Signor Presidente, ringrazio i senatori interroganti per aver opportunamente richiamato l'attenzione del Governo sul tema della carenza di organico delle sedi INPS del Veneto, in particolare di quella di Vicenza. Gli atti di sindacato ispettivo trattano il medesimo tema, pertanto fornirò una risposta congiunta. Sul punto sono state acquisite informazioni dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Per quanto riguarda l'erogazione dei servizi da parte della sede INPS di Vicenza, sentita la struttura competente, si evidenzia che non risultano ritardi nelle emissioni dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC); inoltre, la gestione dei certificati di distacco dei lavoratori in Paesi dell'Unione europea rispetta i tempi previsti dalla Carta dei servizi dell'istituto. risulta che non vi siano ritardi significativi nemmeno nelle erogazioni delle prestazioni sociali ai singoli cittadini, come quelle per malattia, maternità e trattamenti previdenziali in generale. Per quanto concerne la chiusura degli sportelli di Thiene e Arzignano, l'INPS rappresenta che la carenza del personale, unitamente al diminuito interesse da parte dei Comuni nel proseguire le sinergie logistico-funzionali attivate per ospitare i punti INPS, induce le sedi regionali dell'istituto a ripensare la modalità di presidio del tessuto locale e con esso l'organizzazione del lavoro. I punti INPS sono istituiti al fine di garantire prossimità all'utenza in un contesto di maggiore economicità. Attualmente il punto INPS di Thiene è aperto due giorni a settimana e quello di Arzignano un giorno a settimana. L'apertura di entrambe le strutture è assicurata dal personale di missione proveniente dalla direzione provinciale di Vicenza e dall'agenzia di Schio. Riguardo al dimensionamento del personale, INPS evidenzia che il problema delle carenze di organico non è limitato soltanto al Veneto, ma è diffuso in diverse Regioni. Di conseguenza, l'istituto ha indetto nel 2021 un concorso pubblico per 1.858 posti di consulente di protezione sociale. L'espletamento del detto concorso ha consentito di assumere 4.700 nuove unità di personale. La direzione provinciale di Vicenza, con 47 nuove assunzioni, ha visto il trasferimento di tre unità fuori Regione e la cessazione per dimissioni di tre dipendenti. L'istituto ha preso atto, pertanto, della criticità rilevata e ha messo in atto tutte le iniziative del caso, quale il ricorso, mediante appositi avvisi pubblici, al reclutamento di personale in assegnazione temporanea in posizione di comando. A tal proposito si fa presente che attualmente prestano servizio in assegnazione temporanea in posizione di comando presso le strutture INPS del Veneto 30 unità di personale. Nello specifico, presso la direzione provinciale di Vicenza sono attivi sette comandi di personale con profilo amministrativo. Da ultimo, con determinazione del commissario straordinario n. 31 del 26 marzo 2024, l'istituto ha avviato cinque procedure di mobilità rivolte al personale in assegnazione temporanea in posizione di comando presso l'istituto da almeno un anno. Si assicura pertanto che l'istituto sta svolgendo tutte le attività necessarie alla gestione delle carenze di organico in atto nei diversi territori regionali, mediante l'utilizzo delle varie leve gestionali a disposizione e che si terrà conto delle criticità specificamente segnalate in relazione alla Regione Veneto. Inoltre, rinsaldando la volontà di confermare la presenza dell'istituto sul territorio e di non arretrare, è in corso una riflessione allo scopo di individuare ed attuare misure che consentano di superare le problematiche in ordine di organico. Concludo assicurando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a monitorare la situazione e a sostenere tutte le iniziative assunte dall'istituto affinché siano sempre garantiti i diritti dei cittadini.

non possiamo ritenerci in alcun modo soddisfatti; anzi, al contrario, per il tenore della sua risposta, non possiamo che essere ulteriormente preoccupati, perché non mi pare si vedano in tempi rapidi delle soluzioni che possano risolvere il problema del sottodimensionamento delle sedi INPS del Veneto, in particolare di quella di Vicenza. Credo che le nostre preoccupazioni saranno anche quelle delle istituzioni locali, che lei ha citato, del Comune di Vicenza, degli altri Comuni e naturalmente delle imprese e dei cittadini di tutto quel territorio. Penso anche che le procedure concorsuali di cui lei ha parlato non siano sufficienti ad affrontare il problema di assunzioni che siano in grado di rispondere alle esigenze del Veneto e nemmeno la strada degli interpelli è in grado di risolvere quella carenza di personale, anche per l'alto fabbisogno esistente che rimane insoddisfatto. Le vorrei anche dire che la chiusura delle sedi di Thiene e di Arzignano ed il loro presidio molto ristretto è un grave errore, perché ciò che fa dell'INPS, che - ricordiamolo - è un istituto pubblico di *welfare*, l'istituto pubblico più importante d'Europa è, oltre alla capacità di garantire un servizio adeguato, la sua capillarità sul territorio. Ora lei, nella sua risposta, si è appellato a una serie di dati statistici rispetto all'erogazione dei servizi, ma le ricordo che esiste una necessità reale quotidiana che evidenzia chiaramente le difficoltà di cui parliamo e di cui, come parlamentari, peraltro non solo della mia parte politica, siamo stati messi a conoscenza da parte delle istituzioni Lei sa bene, poi, che il Veneto è una delle Regioni più dinamiche d'Europa dal punto di vista economico e sociale, richiede infrastrutture immateriali e materiali che siano in grado di sostenere tale dinamismo e tale vitalità e l'INPS è senza dubbio una di queste infrastrutture sociali. dunque, che il Governo dovrebbe valutare con maggiore attenzione l'impatto che l'INPS, questa importante infrastruttura sociale, può avere nel tessuto economico e sociale di ogni parte del nostro Paese e di una Regione come il Veneto in modo particolare. Credo sia necessario anche valutare l'ipotesi, l'ipotesi, signor Sottosegretario, di indire concorsi anche di carattere regionale - questo non ha niente a che fare, come ben si sa, con l'autonomia differenziata, ma è una questione che è stata già posta in evidenza nel passato - per chi risiede in Veneto,

connessa a quello di cui stiamo parlando: chi vince un concorso pubblico, soprattutto all'inizio, anche all'INPS o nel mondo della scuola, ha uno stipendio abbastanza modesto e spesso per chi proviene da altre Regioni il costo della casa si fa sentire e assorbe gran parte della retribuzione. Sarebbe quindi opportuno provare a sperimentare concorsi di carattere regionale e anche un confronto tra le istituzioni per trovare soluzioni abitative che possano rispondere a tale esigenza, perché il costo della vita e la disponibilità di alloggi è una priorità che non può essere ignorata. Per tali ragioni che il Governo debba continuare a prestare la massima attenzione alla questione e lavorare seriamente per superare questo *vulnus* nella provincia di Vicenza e per risolvere la questione

Signor Presidente, sono un po' in imbarazzo con il Sottosegretario, perché, nonostante sia un componente della maggioranza che sostiene questo Governo, devo dichiararmi insoddisfatto della sua risposta.

po' la questione. La provincia di Vicenza non è una provincia qualsiasi, ma è la prima in Italia per produzione industriale *pro capite*. Noi, come produzione industriale *pro capite*, siamo terzi in assoluto, dopo Milano e Torino, che hanno una popolazione molto superiore alla nostra. Siamo la prima Provincia per quanto riguarda Confartigianato Italia. Abbiamo un tessuto industriale straordinariamente fecondo, imprese che esportano in tutto il mondo. Stando ai dati 2019, ogni cittadino di Vicenza esportava un fatturato di 22.000 euro, compresi il sottoscritto, che fa politica e non esporta nulla, e i bambini. Quindi, stiamo parlando di una realtà particolare, votata all'attività industriale. Elenco alcuni dati che non risultano dalla sua risposta. Nel 2020, presso la sede INPS di Vicenza, vi era un organico di 220 persone: oggi sono 184. da solo, ci dice come in questo periodo ci sia stato un regresso e come questo abbia comportato anche carenze nell'erogazione dei servizi. Credo che sia del tutto plausibile.

è sicuramente un dato che non può essere considerato accettabile. Sono rimasto anche molto sorpreso del fatto che la chiusura delle sedi di Arzignano e di Thiene, secondo la sua risposta, sarebbe dovuta a scarso interesse da parte dei Comuni interessati. Io le dico che la mia interrogazione, in particolare, è stata sollecitata dal sindaco di Thiene, Giampi Michelusi, il quale mi ha fatto presente questa situazione. Pertanto, tenderei ad escludere che ci sia disinteresse da parte dei Comuni o mancata assistenza. Credo che il problema nasca da queste carenze di organico, del tutto inaccettabili. Io auspico e spero che vi si possa porre rimedio. Vi è il problema, sollevato anche dal collega Martella, degli stipendi, che probabilmente per certe mansioni sono troppo bassi, soprattutto se i vincitori di concorso vengono da altre Regioni meno fortunate del Veneto. Questo non vale solo per i dipendenti INPS, ma vale per i cancellieri in tribunale e vale per gli insegnanti. È necessario ovviare a questo problema e sarà un dato normativo sul quale dovremo lavorare. Innanzitutto, vi è bisogno di concorsi regionali e poi di alloggi con dei prezzi calmierati. Altrimenti, le persone vincono il concorso, arrivano a Vicenza, restano il tempo minimo minimo previsto dalla normativa e poi, quando possono, tornano a casa. Quindi, io non posso che ribadire che la risposta non mi pare in linea con le necessità che i diversi

Presidente, noi, invece, siamo qui a ringraziare il sottosegretario Durigon, che per il Ministero del lavoro è venuto qui a rispondere a un'importante interrogazione, riguardante un preciso contesto territoriale. Già il fatto di essere oggi qui, a dare una risposta per certi versi difficile, significa ribadire e confermare l'interesse di questo Governo, non solo per le questioni che riguardano l'intero territorio nazionale, ma anche e soprattutto i temi territoriali. Noi andiamo a leggere la risposta del Ministero, soprattutto sulle parti conclusive, dove vi è un chiaro impegno a monitorare, verificare, migliorare una situazione quale quella rappresentata dalla provincia di Vicenza. Come è stato illustrato anche dai colleghi, la Provincia di Vicenza non è una provincia minoritaria, non è una Provincia

ci stiamo adoperando tutti per far sì che Vicenza meriti l'attenzione del Governo e delle istituzioni per quello che sa fare e produrre. Uno dei temi è quello dell'INPS, ma ve ne sono anche altri.

un futuro riconoscimento di spazi di autonomia per le Regioni e della possibilità che vi siano anche dei concorsi regionali;

da difficoltà sicuramente che, come è stato ben sottolineato dai colleghi, appartengono ad un periodo precedente

parliamo di una Provincia economicamente importante: possiamo definirla una locomotiva del territorio nazionale dal punto di vista del tessuto industriale, ma anche sociale e non solo economico, e i disagi che

almeno momentaneamente quello che ancora non si è in grado di fare con un concorso nazionale, che - lo ripeto - era previsto entro il 2024. Voglio sollevare anche io la questione dei non solo per i cittadini e le imprese, ma anche per gli stessi operatori del settore e le persone che ci lavorano, a cui va il nostro ringraziamento. L'INPS è infatti un istituto molto importante e attivo sul nostro territorio, un punto di riferimento e un'infrastruttura sociale importante,

per avvicinarsi alla Regione di origine in quanto con stipendi così bassi non possono far fronte a tutto ciò che deriva dal vivere in un territorio economicamente importante. Per tutte queste ragioni, mi dichiaro insoddisfatta della risposta.

Signor Presidente, onorevoli senatori, nei mesi scorsi il Ministero dell'interno ha posto in essere diverse iniziative volte a superare le criticità connesse alle tempistiche di rilascio dei passaporti che, come ricordato dall'onorevole interrogante, sono riconducibili a un aumento esponenziale e ravvicinato del numero di istanze di rilascio che si è registrato a seguito di diversi fattori, tra i quali la Brexit e la fine delle restrizioni connesse al Covid. Al fine di mitigare i disagi dell'utenza, sono stati progressivamente attuati interventi di carattere organizzativo (dall'aumento presso le Questure del numero degli sportelli per la ricezione delle istanze, all'ampliamento dei tempi di apertura, fino all'organizzazione di aperture straordinarie in giorni festivi o prefestivi), con il conseguente potenziamento del personale impiegato. Sempre al fine di migliorare il servizio, dal mese di marzo di quest'anno il sistema di prenotazione degli appuntamenti Agenda online è stato implementato con apposita sezione, cosiddetta agenda prioritaria, che consente la rapida gestione delle istanze per coloro che hanno necessità di partire con urgenza per motivi di studio, lavoro, salute o turismo. Per agevolare l'utenza nelle città metropolitana di Torino, Milano e Napoli si è altresì passati a un sistema di emissione dei passaporti centralizzato presso la Questura, con l'emissione diretta da parte dei commissariati di pubblica sicurezza competenti a ricevere le istanze Lo straordinario impegno profuso ha consentito di raggiungere risultati positivi. Infatti, quest'anno - dal mese di gennaio a oggi - sono stati emessi più di 2 milioni e 170.000 passaporti, a fronte di 1,9 milioni rilasciati nello stesso periodo del 2023. Questi risultati, come accennato, sono il frutto di un notevole sforzo organizzativo richiesto alle Questure, dagli interventi di potenziamento delle risorse umane e strumentali a disposizione degli uffici, alla ristrutturazione del sistema di prenotazione *on line*. Un ulteriore e decisivo contributo per rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini è rappresentato dal progetto Polis, che consente di richiedere e rinnovare il passaporto direttamente agli sportelli delle Poste Italiane senza doversi recare in Questura, con la possibilità di ricevere il documento a domicilio. Il Governo, dal marzo scorso, ha dato avvio al progetto e lo sta progressivamente estendendo sul territorio nazionale, con l'attuale coinvolgimento di 213 sportelli dislocati in altrettanti Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Dal mese di luglio è consentita anche l'accettazione delle istanze di rilascio del passaporto a favore dei minorenni, per i quali non sussistono provvedimenti giudiziari che dispongano in ordine alla responsabilità genitoriale o tutoria. Infine, aggiungo che lo scorso mese di giugno è stata siglata una convenzione tra il Ministero dell'interno e Poste Italiane che consente di estendere la modalità di presentazione delle istanze presso gli uffici postali anche nei centri urbani con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Il servizio, che allo stato coinvolge sperimentalmente le città di Roma, Milano, Bologna, Cagliari e Verona, sarà progressivamente esteso all'intero territorio nazionale. Le iniziative illustrate vanno quindi nell'auspicata direzione della semplificazione procedurale e dell'efficientamento complessivo del sistema. In tal senso si sono registrati apprezzamenti sia da parte dei cittadini che delle organizzazioni del comparto turistico. Da ultimo, si assicura che l'amministrazione continuerà a monitorare la situazione affinché il servizio di rilascio dei passaporti avvenga con la massima celerità su tutto il territorio nazionale. [DE

un intervento importante in questi mesi da parte del Governo su un tema che indubbiamente rappresenta un elemento fondamentale per l'esercizio del diritto dei cittadini di

situazioni più urgenti. Sono altresì fondamentali l'accordo e il lavoro fatto insieme a Poste Italiane da parte del Ministero dell'interno sia con il progetto Polis legato ai piccoli Comuni e di fatto già attivo, sia

Signor Presidente, ringrazio i senatori interroganti per il quesito posto, in merito al quale è necessario richiamare sinteticamente i punti salienti della vicenda. Innanzitutto occorre rammentare all'Assemblea che il Ministero della cultura si è assunto la responsabilità di promuovere direttamente, per la prima volta, la candidatura nella lista del patrimonio mondiale della via Appia Regina Viarum. Lo ha fatto per due motivi; prima di tutto perché la via Appia costituisce una testimonianza straordinaria della civiltà romana, che racconta splendidamente la nostra storia e la nostra identità, come valore eccezionale per tutta l'umanità. Per altro verso si trattava di una candidatura complessa alla luce dell'estensione del percorso e dell'esigenza che ciascuna componente proposta rispondesse rigidi parametri dettati dall'UNESCO. È stato perciò realizzato un rigoroso lavoro scientifico di selezione delle componenti del sito seriale, con la consulenza di una commissione scientifica formata da eminenti personalità della cultura e di un comitato tecnico che ha coordinato i lavori di formulazione del *dossier* di candidatura. Al termine di un lungo processo partecipativo a cui hanno collaborato 4 Regioni, 13 tra Province e città metropolitane e oltre 70 Comuni, è stata formulata la proposta di iscrizione nella lista del patrimonio mondiale di un sito seriale, composto da 22 componenti, tutte a nostro avviso pienamente titolate ad essere riconosciute di eccezionale valore universale secondo i canoni della Convenzione per il patrimonio mondiale. Una volta presentata, il Ministero della cultura, in raccordo con la Farnesina e con la Rappresentanza permanente d'Italia all'UNESCO, ha seguito ogni passaggio del lungo e approfondito percorso di valutazione della candidatura. In particolare, ha mantenuto un'interlocuzione costante con il Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti, organo tecnico-consultivo dell'UNESCO, denominato ICOMOS. Con il sostegno del Ministero l'organo ha effettuato, dal 10 al 30 settembre 2023, una missione di valutazione che ha toccato ciascuna delle richiamate 22 componenti del sito candidato. A seguito di detta missione è pervenuta la richiesta dell'ICOMOS di ulteriori informazioni, alla quale questo Dicastero ha fornito un dettagliato riscontro, sempre con il supporto del Comitato tecnico-scientifico. Successivamente, una delegazione composta da rappresentanti del Ministero della cultura e del Comitato tecnico-scientifico ha partecipato a Parigi al *panel* di confronto che, come da prassi, ha rappresentato un momento di interlocuzione per discutere criticità e fornire chiarimenti. In questa occasione l'ICOMOS si è complimentato per la qualità del *dossier* presentato, a fronte di una candidatura estremamente articolata. A seguito della trasmissione da parte dell'ICOMOS del rapporto intermedio di valutazione, l'ufficio competente del Ministero ha fornito puntualmente i chiarimenti richiesti, recependo nella documentazione di candidatura anche i suggerimenti forniti dal medesimo ICOMOS. Nel giugno 2024 ICOMOS ha formalizzato la sua positiva raccomandazione all'iscrizione della via Appia nella lista del patrimonio mondiale, con l'esclusione di tre delle 22 componenti proposte. Nel caso dei tratti 3 (comprendente i Comuni di Genzano, Nemi, Lanuvio e Velletri) e 4 (Latina, Cisterna di Latina, Norma, Sermoneta, Sezze, Pontinia) l'esclusione è stata giustificata sulla base della non perfetta connessione con il tracciato viario principale, contenendo delle deviazioni da esso, in particolare le deviazioni verso Lanuvio e Norba. Nel caso invece della componente 15 (Altamura, Santeramo in Colle, Matera, Laterza e Castellaneta) ICOMOS ha invece giudicato carenti le condizioni di autenticità e di integrità del tratto. La posizione dell'organo tecnico-consultivo, in particolare quando, nel formulare la raccomandazione, si esprime comunque in modo favorevole all'iscrizione (come è stato in questo caso), influenza in maniera determinante l'orientamento dei membri del Comitato del patrimonio, chiamati a decidere sulla proposta di candidatura. Questo Ministero, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha perciò ritenuto opportuno prendere atto della raccomandazione, in modo tale da non mettere a rischio l'iscrizione del sito via Appia Regina Viarum nella sessione 2024 del Comitato. Ha tuttavia immediatamente avviato un'interlocuzione con i vertici di ICOMOS per esprimere contrarietà in merito alle valutazioni contenute nel rapporto, che non prendono in considerazione gli articolati argomenti tecnici presentati a sostegno dell'iscrizione delle tre componenti, soprattutto il dato storico-culturale che le vede parti qualificanti ed imprescindibili dell'Appia antica. Questo Dicastero intende intraprendere, con determinazione e in collaborazione con il MAECI, i Comuni e le comunità interessate, ogni possibile iniziativa volta ad ottenere dall'UNESCO, nel più breve tempo possibile, l'ampliamento dell'area iscritta nella lista del patrimonio mondiale, conformemente all'originaria candidatura. A questo fine ho convocato per il prossimo 26 settembre una prima riunione con gli amministratori locali interessati, per programmare le attività necessarie ad elaborare una richiesta di estensione del sito della via Appia alle componenti escluse nella decisione finale del Comitato del patrimonio mondiale. Si precisa inoltre che per questo Ministero e per il Governo i Comuni che hanno partecipato all'elaborazione della candidatura e che hanno sottoscritto nel gennaio 2023 il relativo protocollo d'intesa sono a pieno titolo parte del progetto collettivo di valorizzazione della via Appia. Ciò vuol dire che le amministrazioni interessate saranno coinvolte dal Ministero della cultura nelle iniziative di tutela, conservazione e valorizzazione del percorso e verranno associate ai meccanismi di attuazione del piano di gestione del sito, nel quale, tra l'altro, sono già contemplate anche ai fini della destinazione di risorse finanziarie. Lavoreremo con tutta la comunità di enti che hanno promosso la candidatura del sito "Via Appia. Regina Viarum", affinché il prestigioso riconoscimento ottenuto con l'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale produca opportunità di sviluppo socioeconomico per i territori e per le comunità che li abitano.

grande obiettivo ottenuto ed è stato importante che il Ministero abbia lavorato insieme agli enti locali e alle Regioni interessati, perché stiamo parlando - come dice Paolo Rumiz - della madre di tutte le vie, dimenticata però in secoli di incuria e ignoranza.

del 2016, il ministro Franceschini istituì un tavolo proprio per valorizzare il percorso della grande diagonale del Mediterraneo. È un monumento lineare, un cammino laico, un cammino laico, che non ha nulla da invidiare alla via Francigena o ad altri cammini, e comunque sappiamo che un cammino è sempre anche un cammino dell'anima. È davvero un sito incredibile e una strada

1.823 ettari importanti per la storia di questa strada. Penso alla provincia di Roma, ma anche alla provincia di Latina: penso a Cisterna di Latina e a che cosa significa quel sito. Sono paesaggi naturali e antropizzati, paesaggi importanti. Penso anche alle Province di Matera, di Matera, di Taranto e di Bari. Forse una certa fretta a un certo punto di chiudere ci ha fatto perdere l'occasione di ottenere il riconoscimento dell'intera strada, ma è molto importante capire quali sono gli atti che il Ministero metterà in campo assieme ai Comuni. Sappiamo della riunione. È molto importante vedere atti concreti, perché ci possa essere il riconoscimento e soprattutto, visto che quei Comuni hanno partecipato e la via è un *unicum*,

il percorso non escludano quei Comuni che oggi non sono compresi nel riconoscimento del sito. Questo è molto importante per tenere compattamente insieme il percorso dell'Appia, anche perché

Si è così concluso lo svolgimento delle interrogazioni. Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il *question time*. *(La seduta, sospesa

finestra"). Comunico che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 è convocata mercoledì 18 settembre alle ore 8,30 presso la sede di Palazzo San Macuto per procedere alla propria costituzione. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'istruzione e del merito.

fin dall'inizio del suo mandato, il Ministro in indirizzo ha avviato un'intensa azione politica che pone al centro la stabilizzazione dei Balcani occidentali, la loro prospettiva europea e una maggiore presenza dell'Italia e delle imprese italiane nella regione; l'ultimo biennio ha visto importanti traguardi dal punto di vista del percorso di adesione europea dei Balcani occidentali, a cui l'Italia ha contribuito attivamente; diverse sono le iniziative lanciate per sviluppare ed approfondire i legami politici, economici e sociali tra il nostro Paese e i Paesi della regione, tanto a livello bilaterale quanto regionale - mi consenta di dirlo - a cui ha contribuito anche la Commissione esteri e difesa del Senato. citare la recente visita a Podgorica e a Skopje del 10 settembre 2024, in cui il Ministro interrogato ha ribadito l'impegno dell'Italia e la sua volontà di continuare a sostenere il percorso di integrazione europea dei Paesi dei Balcani occidentali. quindi di sapere quali ulteriori iniziative abbia intenzione di intraprendere il Ministro per continuare a dare impulso all'azione dell'Italia nei Balcani occidentali, alla cooperazione economica con i Paesi della regione e al loro percorso di integrazione europea. PRESIDENTE.

del nostro Governo. Negli ultimi due anni, l'Italia è tornata ad essere protagonista nella regione attraverso una presenza costante e concreta. Lo confermano le mie recenti visite l'altro ieri in Montenegro e in Macedonia del Nord, con cui ho completato il giro di tutti i Paesi della regione. Negli incontri che ho avuto con i miei interlocutori ho voluto trasmettere un messaggio di forte attenzione dell'Italia sia a livello politico che sul piano economico. È un'area per noi vicina geograficamente e fondamentale sul piano strategico, non dobbiamo lasciare all'influenza di altri Paesi rivali e ostili. Il nostro Governo continua in tutte le sedi a promuovere l'obiettivo della riunificazione dell'Europa. A Bruxelles sto lavorando affinché il *dossier* sia prioritario anche per la nuova Commissione. Abbiamo già pianificato per i prossimi mesi una riunione che vorremmo ospitare a Roma con i Ministri degli esteri dei Paesi balcanici e il prossimo commissario per l'allargamento. A New York tra pochi giorni, a margine di una settimana di alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ci riuniremo con i Paesi della regione per un nuovo incontro del gruppo degli amici dei Balcani insieme ad Austria, Croazia, Grecia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia. Certo, le sfide non mancano, come dimostra, ad esempio, il complesso dialogo tra Serbia e Kosovo. A breve riassumeremo il comando della missione NATO Kosovo Force (KFOR) con il generale Barduani. Siamo orgogliosi del ruolo che svolgono nella regione i nostri militari, che godono dell'ammirazione e del rispetto di entrambe le parti. Il percorso d'integrazione politica va di pari passo con il rafforzamento dei partenariati economici, strumenti importanti per la stabilità e il dialogo. In Montenegro ho partecipato, insieme al Ministro degli esteri, al tavolo energia, con l'ambizioso obiettivo di integrare il mercato dell'energia elettrica montenegrino con quello italiano. Il tema della connettività delle infrastrutture strategiche è infatti fondamentale per avvicinare le due sponde dell'Adriatico e approfondire la cooperazione economica, a partire dal Corridoio 8, sulla base della riunione ministeriale che ho organizzato a Brindisi nei mesi scorsi. In questi anni, ho organizzato incontri con i nostri imprenditori per rafforzare la presenza economica italiana nella regione e l'internazionalizzazione delle nostre imprese. A Skopje, dove ho avuto modo di incontrare i principali operatori economici italiani, abbiamo deciso di organizzare quanto prima un *business* *forum* anche in Macedonia del Nord con aziende italiane e locali per promuovere gli investimenti. L'integrazione dei Balcani, in conclusione, deve essere una priorità della nuova legislatura europea. La riunificazione dell'Europa - preferisco questo termine a quello di "allargamento" - non potrà infatti dirsi completa senza i Balcani occidentali.

*(M5S)*. Signor Ministro, a gennaio la Corte internazionale di giustizia ha chiesto ad Israele di prevenire atti genocidari nella Striscia di Gaza, mentre nel mese di luglio ha dichiarato illegale l'occupazione dei territori palestinesi da parte di Israele. A maggio di quest'anno la Corte penale internazionale, a mezzo del suo procuratore capo, ha chiesto un mandato d'arresto per il primo ministro Netanyahu e per il Ministro della difesa, ritenendoli responsabili di crimini di guerra e contro l'umanità. Un mese dopo, a giugno, la Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha accusato Israele di crimini di guerra come sterminio, deportazione e tortura. Soltanto pochi giorni fa, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha dichiarato inaccettabile l'uso di armi pesanti in zone densamente abitate, dopo l'ennesimo *raid* israeliano. Ad aprile di quest'anno, una risoluzione del Consiglio dei diritti umani dell'ONU ha chiesto l'embargo globale su tutti i tipi di armi a Tel Aviv, mentre dobbiamo constatare che il Regno Unito ha sospeso decine di licenze e il Governo italiano si è limitato a non rilasciarne di nuove. Soprattutto, dati Istat di - dichiarano che, dopo il 7 ottobre 2023, il nostro Paese ha mandato ad Israele armi per un valore di 4,6 milioni di euro. Infine, il Ministro israeliano dell'energia e delle infrastrutture nell'ottobre del 2023 ha annunciato l'assegnazione ad ENI di licenze di esplorazione di giacimenti di gas al al largo delle coste di Gaza, un territorio che per il 62 per cento, in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, è palestinese. Per questo quattro associazioni palestinesi per i diritti umani hanno inviato avviso ad ENI di non intraprendere le suddette attività. Sulla base di queste premesse, signor Ministro, le chiedo: intende richiamare l'ambasciatore italiano a Tel Aviv in segno di protesta contro le violazioni del diritto internazionale e i crimini di guerra commessi da Israele a Gaza? Il nostro Paese intende sospendere le esportazioni di armi italiane verso Israele, come richiesto

Signora Presidente, in Medio Oriente la posizione dell'Italia è sempre la stessa: lavoriamo per la pace, perché ci sia il cessate il fuoco a Gaza, ci sia la liberazione degli ostaggi, sia rafforzato l'accesso umanitario, si possa pianificare un percorso che porti a uno Stato palestinese che riconosca Israele e sia riconosciuto da Israele, e quindi due popoli e due Stati. Bisogna allentare la tensione con l'Iran e in tutta la regione bisogna impedire che ci sia una *escalation* che provochi un conflitto più ampio. Stiamo lavorando proprio per scongiurare questo pericolo come Presidenza G7, insieme all'Unione europea, ma soprattutto in costante contatto con i nostri *partner* dell'area mediorientale. Tutti ci riconoscono l'autorevolezza di chi ha mantenuto sin dall'inizio della crisi una posizione seria ed equilibrata ed apprezzano il ruolo di ponte che stiamo svolgendo in questa crisi. Non è un caso che il nuovo primo ministro palestinese Mohammad Mustafa abbia scelto di venire a Roma in occasione della sua prima missione all'estero. Ora più che mai occorre sostenere gli sforzi di mediazione che gli Stati Uniti stanno compiendo insieme all'Egitto e al Qatar per il raggiungimento di un accordo tra le parti. Nelle ultime settimane ho continuato ad essere in contatto con i Ministri degli esteri della regione e ho reiterato a tutti gli attori coinvolti appelli al dialogo e alla moderazione, Israele e Iran inclusi; ho ricevuto il loro apprezzamento per la nostra iniziativa Food for Gaza. Sulla questione dell'esportazione di armi verso Israele - come ho già avuto modo di riferire più volte in Parlamento - l'approccio del Governo è sempre stato improntato alla massima cautela. Ribadisco che dal 7 ottobre non sono state concesse nuove autorizzazioni a esportare armi verso Israele. La sospensione prosegue tuttora. È una posizione cauta ed equilibrata che è stata apprezzata anche dei principali organismi internazionali in materia. Sull'assegnazione di blocchi esplorativi *offshore* ad ENI da parte di Israele, confermo che si tratta di una gara internazionale a cui ENI ha preso parte con altri due operatori, nel rispetto delle regole. Da quanto riferisce ENI, il contratto è ancora in fase di negoziazione. Il consorzio perciò non ha alcuna titolarità sull'area né sono in corso operazioni che avrebbero comunque natura esplorativa. Non vi è dunque, al momento, alcuno sfruttamento di risorse. Tanto Israele quanto l'Autorità nazionale palestinese hanno diritto a sfruttare le risorse del mare nel rispetto delle norme internazionali, e anche in questo la strada maestra non può che essere il negoziato per raggiungere un accordo equo che tuteli i diritti di ciascuno. In questa fase particolarmente delicata è fondamentale mantenere ed espandere tutti i canali di dialogo per allentare le tensioni e interrompere la spirale di violenza che rischia di innescare un conflitto in tutta la regione.

il nostro giudizio non può che essere negativo su tutta la linea. Con le sue risposte-non risposte lei ha dimostrato che questo Governo, al di là delle vuote parole, dice di lavorare per la pace, ma poi in realtà continua a scegliere di sostenere politicamente, economicamente e militarmente il criminale Governo di Netanyahu e, quindi, ad essere complice del disumano sterminio del popolo palestinese. Anche oggi ci sono state notizie di bombardamenti su edifici che dovrebbero essere sicuri (scuole, ospedali, campi profughi) e c'è la morte di rappresentanti dell'Agenzia dell'ONU per la protezione del popolo palestinese. Per noi è inaccettabile pensare che tra le bombe che cadono sulla testa della popolazione inerme e che uccidono civili, donne, bambini e ammalati ci sia materiale bellico che arriva dal nostro Paese. Per noi è inaccettabile sentire i medici che tornano dalle missioni umanitarie dire che in media quattro bambini al giorno arrivano con ferite da arma da fuoco alla testa, perché pare siano come dei bersagli mobili, delle vittime predestinate dei cecchini israeliani. Tutto questo non lo tolleriamo e se voi, come rappresentanti di questo Paese e come Governo italiano, non fate niente, siete complici

Signor Presidente, come Gruppo Partito Democratico conosciamo la complessità del rapporto con l'Azerbaijan sotto più di una dimensione. *Partner* strategico dal punto di vista energetico, è sicuramente un Paese in prospettiva fondamentale per la stabilizzazione dell'area. Allo stesso tempo, a un Paese con cui abbiamo una *partnership* strategica non possiamo non dire quando ci sono alcune cose che non funzionano, soprattutto nel mancato rispetto dei diritti umani. Ciò è quanto è stato fatto presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europea alcuni parlamentari (anzi, la maggioranza dei parlamentari trasversalmente a tutti i gruppi politici) e, in particolare, cinque parlamentari italiani: tre del Senato (le senatrici Zampa e Floridia e il senatore Verducci) e i deputati Fassino e Orlando. Si è arrivati a votare e a non ratificare le credenziali delle delegazioni dell'Azerbaijan dopo un anno molto complicato che ha visto un conflitto nel Nagorno Karabakh, ma soprattutto un un lavoro molto attento del Consiglio d'Europa e dell'Assemblea parlamentare nell'andare a stigmatizzare alcune cose che non funzionano in quel Paese: oltre 200 prigionieri politici, la mancanza della garanzia dei diritti delle minoranze la garanzia dei più elementari diritti civili nel Nagorno Karabakh. Sono tutte cose che il Ministro degli affari esteri conosce molto bene per la sua esperienza nei diversi ruoli che ha ricoperto. Purtroppo quella mancata ratifica è stata solo una conseguenza del fatto che non si è mai risposto alle osservazioni del Consiglio d'Europa e soprattutto non sono stati fatti entrare i tre *rapporteur* sulla situazione dell'Azerbaijan ed è stata negata la possibilità alla delegazione dei parlamentari presso il Consiglio d'Europa di tutti i gruppi politici. Ricordo che uno dei principali *rapporteur* è addirittura del gruppo dei conservatori europei, della destra europea inglese. A questo punto è stato inevitabile votare a larghissima maggioranza la mancata ratifica. Purtroppo c'è stata una reazione spropositata da parte dell'Azerbaijan: le 76 persone che avevano votato sono state dichiarate persone non grate e non sono potute entrare in Azerbaijan e non c'è stata la delegazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a verificare le elezioni. Purtroppo il 5 settembre c'è stato un incontro della presidente del Consiglio Meloni, con accordi importanti siglati con l'Azerbaijan. Tuttavia, non abbiamo visto, né sentito esponenti del Governo prendere posizione in maniera netta a tutela e a difesa dei difesa dei parlamentari delle nostre Assemblee. Questo è ancor più grave perché sono parlamentari dell'opposizione. Ci saremmo aspettati una parola chiara da parte del Ministro degli affari esteri o della Presidente del Consiglio.

Presidente, mi permetta di protestare perché durante il precedente *question time* una senatrice si è rivolta a me in quanto segretario del partito, attaccandomi per alcune scelte fatte alla Camera dei deputati. Siccome non posso rispondere dai banchi del Governo, perché sono qui in veste di Ministro degli affari esteri, mi sembra veramente un po' maramaldesca questa posizione di poco coraggio. Sono comunque pronto a confrontarmi, ma vedo che la senatrice è scappata, non è più presente in quest'Aula. Devo protestare, però, signor Presidente, perché non è questo il modo corretto di comportarsi durante un *question time*. Se deve fare un dibattito politico, lo fa quando c'è qualcuno che può rispondere e non quando c'è qualcuno che non può rispondere perché qui in veste di Ministro. Non ho risposto nel merito. Signor Presidente, mi rivolgo a lei perché non mi posso rivolgere agli onorevoli senatori, ma è stata molto scorretta. Ribadisco che questo atteggiamento è stato scorretto nei confronti del Governo.

Lo scorso 24 gennaio l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha deciso di non ratificare le credenziali presentate dalla delegazione parlamentare dell'Azerbaigian. Ciò ha determinato di fatto la sua sospensione dall'Assemblea per l'anno in corso. Il confronto tra Azerbaigian e Consiglio d'Europa si è ulteriormente inasprito lo scorso 2 settembre, quando Baku ha dichiarato come persone non grate 76 parlamentari che avevano votato a favore della risoluzione; tra questi, come ricordato dall'interrogante, vi sono anche cinque parlamentari italiani. La decisione di Baku è stata immediatamente criticata dall'Italia in Consiglio d'Europa. Al Comitato dei Ministri dello scorso 3 settembre, su mie istruzioni, il rappresentante permanente italiano è intervenuto per protestare contro la decisione e incoraggiare la pronta ripresa di un dialogo tra l'assemblea parlamentare e l'Azerbaigian. Il 5 settembre, in occasione della visita a Roma del presidente Aliyev, il Presidente del Consiglio ha sollevato la questione durante l'incontro bilaterale a Palazzo Chigi nel contesto delle relazioni tra Baku e l'Europa. La decisone di vietare l'ingresso nel Paese ai cinque parlamentari italiani è stata dunque oggetto di discussione anche al più alto livello. Solleverò nuovamente la questione tra pochi giorni a New York, dove incontrerò il Ministro degli esteri azero, a margine della settimana di alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. L'Italia difende con convinzione il principio dell'inviolabilità delle prerogative parlamentari. Al contempo, sosteniamo un approccio inclusivo volto a favorire il rientro della delegazione azera nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, a condizione di un reale impegno di Baku in tal senso. Il partenariato con l'Azerbaigian rimane ineludibile per favorire la stabilizzazione regionale e il processo di normalizzazione con l'Armenia. Nelle interlocuzioni con entrambe le parti, il Governo ha sempre mantenuto una posizione equilibrata e costruttiva, incoraggiando un'intesa complessiva di pace. L'Azerbaigian è anche un *partner* significativo a livello bilaterale, come testimoniato dai recenti incontri di alto livello del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio con il presidente Aliyev. I nostri rapporti con Baku continueranno a essere improntati a un dialogo franco e costruttivo, anche per incoraggiare un maggiore impegno da parte azera in ambito multilaterale.

soddisfatta o consolata da quello che lei ci ha rivelato poco fa, che però è stato tenuto assolutamente riservato. Mi riferisco al fatto che la presidente Meloni avrebbe fatto cenno, nel corso dell'incontro con il presidente Aliyev, a quanto avvenuto e, cioè, alla *black list*. Delude però profondamente il fatto che il Governo non abbia compreso immediatamente che bisognava dare in qualche modo modo visibilità e contezza di una presa di posizione alla quale avevamo diritto non solo io che sono una dei 76 e i cinque parlamentari, ma credo il Paese e il Parlamento.

a difesa del ruolo che i parlamentari sono chiamati a svolgere nelle sedi internazionali. Io credo che quei cinque parlamentari italiani andrebbero ringraziati da parte del Governo italiano per avere fatto

grazie per averci rivelato che la presidente Meloni ne ha parlato; ci si attende un passo ulteriore importante. il 28 luglio in Venezuela finalmente il popolo si è ribellato alla dittatura e, nonostante le difficoltà imposte dal regime con ogni mezzo di impedire l'accesso degli elettori ai seggi), ha decretato la fine del regime stesso, perché il 70 per cento dei venezuelani ha votato contro Maduro e ha scelto un altro presidente. Come accade in molti regimi, Maduro non ha accettato l'esito delle elezioni e sta reprimendo con ogni mezzo la popolazione e l'opposizione. Non ha risparmiato nessuno e non ha neanche evitato di imprigionare quasi 300 bambini (come a noi risulta). Siamo molto preoccupati per quanto sta avvenendo, non solo perché si tratta e si parla di diritti umani, ma anche perché molti dei nostri connazionali vivono e abitano là. Sappiamo che otto italo-venezuelani sono adesso incarcerati sappiamo che molti altri nostri connazionali e familiari di nostri connazionali hanno subito la stessa sorte, come il portavoce della stessa Corina Machado. Volevamo avere qualche informazione in più in merito allo specifico caso di Americo de Grazia, perché, rapito (non si può usare altro termine) dagli agenti della polizia del regime di Maduro l'8 luglio, supponiamo - e dico supponiamo perché a tutt'oggi non abbiamo la prova né del fatto che sia lì, né del fatto che, ahimè, sia ancora vivo sia detenuto nel carcere "El Helicoide", che è il carcere più duro ed è ritenuto anche un luogo di tortura non solo di Caracas, ma dell'intero Latinoamerica. Siamo molto in apprensione, anche perché negli ultimi giorni non solo non è stato consentito l'accesso ai familiari, ma i secondini questa volta non hanno neanche accettato, nell'ultimo incontro, di dare al supposto detenuto generi di conforto e farmaci. Concludendo, vorrei sapere se lei signor Ministro ha qualche informazione in più

l'attenzione mia e del Governo sulla crisi in Venezuela continua ad essere altissima. La posizione dell'Italia, che ho voluto promuovere anche in ambito G7, forte del mandato unitario ricevuto dal Parlamento, è chiara: l'esito elettorale proclamato dalle autorità venezuelane non ha alcuna legittimità. Fin dall'inizio della crisi in Venezuela la tutela degli oltre 160.000 connazionali presenti nel Paese resta una priorità del Governo. Su mia indicazione al Ministero degli esteri è stata costituita, da inizio agosto, una *task force* permanente per monitorare gli sviluppi nel Paese. In questo contesto vengono affrontati i temi legati all'emergenza e vagliate le iniziative a tutela dei cittadini italiani. In Venezuela l'ambasciata, il consolato generale a Caracas e il consolato a Maracaibo continuano a lavorare senza sosta per assistere i concittadini residenti nel Paese. La nostra attenzione è rivolta soprattutto a chi è privato della libertà personale. Sulla base delle richieste di assistenza pervenute dai familiari dall'inizio della crisi, risultano - come diceva l'onorevole interrogante - attualmente detenuti otto connazionali, tutti doppi cittadini italo-venezuelani. Tra questi vi è Americo de Grazia, ex deputato dell'opposizione all'Assemblea nazionale, che nel 2019 era stato temporaneamente ospitato nella residenza dell'ambasciatore italiano a Caracas, prima di poter lasciare una prima volta il Paese grazie anche ai buoni uffici del presidente Casini, membro di questa Assemblea. Il connazionale nel frattempo, ritornato in Venezuela, è scomparso il 7 agosto dopo essersi recato in una clinica per accertamenti medici. Secondo quanto riportato dai familiari, si troverebbe recluso presso «El Helicoide», un noto carcere militare di Caracas, con l'accusa di incitamento all'odio. Su mia indicazione, l'ambasciata d'Italia a Caracas sta seguendo il caso con il massimo impegno, mantenendo stretti e costanti contatti con i familiari e con i legali del signor De Grazia. Abbiamo chiesto fin da subito l'autorizzazione a effettuare una visita consolare al connazionale. L'ambasciata ha condannato con fermezza le misure detentive adottate nei confronti del signor De Grazia, come di tutti i nostri cittadini, ed espresso forte preoccupazione per la compressione dei loro diritti di difesa. Ci siamo anche associati al passo promosso dalla delegazione dell'Unione europea in Venezuela per invocare la scarcerazione di tutti i detenuti politici con cittadinanza europea, ivi incluso il signor De Grazia. Ferma condanna è stata espressa anche all'incaricata d'affari venezuelana, appositamente convocata alla Farnesina. Le è stata rappresentata la ferma aspettativa che vengano rilasciati i connazionali sottoposti a misure detentive e sia garantito loro un adeguato accesso alla protezione consolare. Continuiamo a monitorare con la massima attenzione l'evoluzione della situazione e a prestare ogni possibile assistenza ai connazionali e ai loro familiari, anche attraverso una costante pressione sulle autorità di Caracas. Voglio ribadirlo anche qui nell'Aula del Senato, che segue da vicino questa vicenda: il popolo venezuelano, così legato all'Italia da vincoli storici e di sangue, merita un futuro di democrazia e di libertà. Continuiamo a lavorare per questo obiettivo con convinzione e determinazione.

conosco essere stato l'interessamento e l'impegno della Farnesina e della *task force* immediatamente organizzata, sempre efficace, efficiente e disponibile nei nostri confronti, ma anche e soprattutto perché l'Italia, sin da subito, ha saputo schierarsi dalla parte della verità e della democrazia senza alcuna ambiguità ed è stato membro proponitore, insieme agli altri membri del G7, di una risoluzione sul Venezuela. Quindi, noi fin da subito, col Governo Meloni, ci siamo schierati dalla parte del popolo e questa, secondo me, è stata la cosa più importante. Colgo l'occasione anche per ringraziare da questa parte del mondo tutti i venezuelani che hanno svolto il rito del voto. Molte volte qua in Italia, purtroppo, ci dimentichiamo il valore e il significato dell'andare a votare. Nonostante tutte le difficoltà, ringrazio tutti coloro che sono rimasti, a differenza degli 8 milioni di venezuelani che purtroppo hanno preferito andare via. Concludo dicendo che, come italiani e come Paese democratico, non possiamo che continuare a fare pressione internazionale per stare sempre dalla parte del popolo, della verità e della democrazia.

Signor Presidente, colleghi, ministro Salvini, la sicurezza stradale è un tema dell'agenda politica che non può avere colori di appartenenza. Credo che su questo punto possiamo essere tutti d'accordo: tutti d'accordo: gli autovelox, oltre 11.000 in tutta Italia, da Nord a Sud, sono uno strumento della sicurezza stradale. Sottopongo oggi alla sua attenzione, signor Ministro, una questione che mi è stata più volte richiesta da sindaci, sia di centrodestra che di centrosinistra, oltre chiaramente da molti cittadini. L'ordinanza della Corte di cassazione n. 10505 del 18 aprile 2024 afferma che, per il legittimo utilizzo dell'autovelox, non è sufficiente la semplice approvazione, ma è necessario che il dispositivo venga omologato. Approvazione e omologazione, in estrema sintesi, solo due procedimenti distinti. A seguito di questa ordinanza, purtroppo, si è creata una situazione di incertezza amministrativa che oggi sottopongo all'attenzione del Dicastero da lei guidato. Infatti, considerando che gli autovelox attualmente in uso sono approvati in forza a un decreto del 2017, ma che nessuno di essi è omologato, si pone un problema di potenziale illegittimità di tutte le sanzioni relative alle violazioni dei limiti di velocità del codice della strada rilevata da quei dispositivi. L'illegittimità delle sanzioni - come è facile immaginare - ha dei riflessi e delle conseguenze molto sentite dai singoli cittadini, da tantissimi sindaci che hanno gli autovelox approvati - come dicevo - ma non omologati. Secondo noi è essenziale porre rimedio a questa situazione di incertezza, definendo in maniera chiara la disciplina sulle modalità di uso degli autovelox, con l'obiettivo - credo condiviso da tutti - di garantire certezza e trasparenza a beneficio di tutti i cittadini *in primis* e di conseguenza di tutti i nostri sindaci, anche alla luce delle indicazioni fornite dal decreto adottato dal Ministero dei trasporti il 12 aprile 2024, concernenti le modalità d'uso dell'autovelox in maniera conforme alle norme previste dal codice della strada e agli obblighi di segnalazione agli utenti della strada stessa. Al signor Ministro presente in Aula, che ringrazio, chiedo pertanto di sapere quali siano le iniziative che il Ministero intende adottare per risolvere le criticità evidenziate in premessa, sanare questo *vulnus* normativo e proseguire nel percorso intrapreso per garantire la sicurezza stradale a tutela dei nostri cittadini e di moltissimi amministratori. trasporti*. Signor Presidente, colleghi senatori, ringrazio per il quesito che si ripete ormai da alcune settimane e che mi consente di fornire chiarimenti su un tema molto sentito, ovviamente, dai cittadini e dai sindaci dopo la sentenza richiamata. Ritengo innanzitutto doveroso precisare che tale decisione riguarda soltanto l'uso dei dispositivi per le violazioni dei limiti di velocità, ma non tutti gli altri, come ad esempio per la rivelazione di ingresso abusivo nelle ZTL o per il passaggio con il semaforo rosso, evidentemente. Tale precisazione è rilevante, perché ricordo che nel disegno di legge di riforma del codice della strada, che il Senato ha già approvato e che conto che la Camera approvi definitivamente entro settembre, è stato inserito un articolo che rimodula le violazioni, che possono essere sanzionate con l'uso di dispositivi senza contestazione immediata. Non mi soffermo sulla decisione, quanto sulle soluzioni che come Ministro ho il dovere di affrontare a stretto giro. Confermo che la messa a terra di tali soluzioni è legata al disegno di legge sulla sicurezza stradale di cui parlavo e aggiungo che lo scorso 3 settembre, quindi pochi giorni fa, ho comunicato direttamente all'ANCI, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, al Ministero dell'interno e al Ministero del *made in Italy*, che sono competenti sul tema autovelox insieme a me, l'intenzione di istituire presso il mio Ministero un tavolo tecnico di settore immediato, concreto ed efficace, per la regolazione delle regole di base per l'omologazione di tutti i dispositivi strumentali, compresi gli autovelox. Il tavolo coinvolgerà tutti gli attori a vario titolo competenti. L'auspicio è che, con il supporto dei tecnici del settore, si possano individuare le nuove regole sull'omologazione per arrivare a una soluzione del problema che abbiamo ereditato. Ribadisco che sul tema servono soluzioni equilibrate, e l'ho ribadito anche ai sindaci. Il mio obiettivo è garantire che gli autovelox siano autorizzati per la sicurezza stradale in chiave di prevenzione e deterrenza e non come ulteriore gabella o tassa, magari su strade a due, tre, quattro corsie, a basso tasso di incidentalità. Ricordo che la stessa linea di equilibrio e di buonsenso stiamo conducendo sulle cosiddette zone a 30 all'ora, che alcuni sindaci stanno applicando. La direttiva che ho firmato prevede che questa fissazione generalizzata dei limiti di velocità inferiori a quelli previsti, quindi le zone a 30 all'ora, venga determinata dove ci sono pericoli o dove sono alti i tassi di incidentalità, motivati su alcune zone della città e non sul 60, 70, 80 per cento della superficie cittadina, come ad esempio accaduto a Bologna. conferma il fatto che i 30 all'ora possano essere un problema anche ambientale, oltre che lavorativo di traffico, in base al recente studio del MIT, non del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di piazza di Porta Pia a Roma, ma del MIT di Boston; quindi autovelox ZTL, limitazioni al traffico e zone a 30 all'ora utilizzate con buonsenso in zone parziali della città e non applicate con ideologia per combattere le auto che - piaccia o non piaccia - a molta gente servono per andare a lavorare.

Signor Ministro, gli organi di polizia dei Comuni lamentano l'impossibilità di accedere alla piattaforma EUCARIS per lo scambio di informazioni sui veicoli con l'Austria, la Germania e anche con l'Olanda. EUCARIS è il sistema digitale di interscambio dei dati di immatricolazione dei veicoli circolanti nei Paesi dell'Unione europea; esso serve alle forze di polizia dei Comuni per risalire ai proprietari delle automobili cui è stata accertata un'infrazione per avviare i procedimenti sanzionatori a loro carico. La disattivazione della piattaforma da parte di Austria, Germania ed Olanda sta privando i Comuni italiani della possibilità di notificare le sanzioni ai veicoli provenienti da quei Paesi. Secondo quanto dichiarato in risposta ad una interrogazione diretta alla Commissione europea, le autorità di quei Paesi avrebbero giustificato tale decisione a seguito dell'individuazione di un uso improprio di dati personali da parte di un'azienda italiana. La commissaria Adina Valean ha parlato di un comportamento illecito persistente, senza specificare però in cosa consisterebbe. Il blocco del sistema di interscambio interessa numerose località turistiche e soprattutto i territori di confine, come l'Alto Adige-Südtirol. Per dare un'idea delle dimensioni del problema, il solo comune di Merano, che conta all'incirca 41.000 abitanti, negli ultimi mesi ha accumulato 4.000 verbali di contravvenzione non notificati, per un importo totale che supera i 230.000 euro. Questa non è solo una discriminazione verso gli automobilisti italiani ai quali viene prontamente contestata ogni infrazione, ma è anche un problema per le casse dei Comuni. Tutto ciò premesso, si chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza dei motivi che hanno portato alla disattivazione di EUCARIS da parte di Austria, Germania e Olanda nei confronti dell'Italia quali iniziative intenda intraprendere, anche in sede europea, per garantire il tempestivo ripristino del sistema.

di Austria, Germania e Olanda. L'automobilista italiano che incorresse in un'infrazione in Austria viene raggiunto dalla multa, come è giusto che sia, in Italia; non vale però il contrario per quelli che dalla Germania, dall'Austria o dall'Olanda vengono in Italia, magari a fare le corse, e poi tornano nel loro Paese. Il problema è in via di soluzione, sostanzialmente quasi immediata. È una questione che stiamo affrontando con la massima determinazione, perché - come si diceva - ha implicazioni dal punto di vista non solo ricordava - ma anche della sicurezza stradale. È inutile che noi rinnoviamo il codice della strada in Italia quando non siamo in grado di garantirlo nei confronti di chi arriva dall'estero. Pertanto, assicurare il rispetto delle norme del codice della strada da parte dei conducenti stranieri quando sono nel nostro Paese rappresenta un un impegno mio e di tutto il Governo. Il sistema di cooperazione che la senatrice interrogante citava ha reso più semplice e automatica l'individuazione di veicoli e conducenti in caso di crimini transfrontalieri, come nel caso - lo ricordiamo - del tragico evento che ha causato la scomparsa del campione italiano di ciclismo Davide Rebellin. Per quanto riguarda la decisione delle autorità olandesi, austriache e tedesche di bloccare lo scambio con l'Italia dei dati di immatricolazione dei veicoli, questa è avvenuta a seguito di problemi tecnici riscontrati sul sistema che abbiamo già risolto, mentre oggi le rispondo. Al riguardo, abbiamo inoltre avviato una costante interlocuzione con i tre Paesi interessati, che ha già portato all'impegno da parte della Germania a ripristinare il sistema di interscambio con l'Italia a partire dal corrente mese di settembre, alla luce dei correttivi che abbiamo messo in atto. Confido che tale impegno con i *memorandum* che stiamo portando avanti venga onorato nei prossimi giorni da parte della Germania e, nel breve periodo, anche da parte di Olanda e Austria nella stessa direzione; appena firmeranno, mi periterò di informare lei e gli altri colleghi dell'avvenuta dell'avvenuta sottoscrizione. In ogni caso, l'argomento è oggetto di discussione a livello europeo, con particolare riferimento alla necessità di revisionare la direttiva integrale del settore, ampliando in particolare le fattispecie di violazioni sanzionabili, il cui numero oggi è ridotto. Sul tema, infatti, la stessa Lega, la mia parte politica, aveva sollevato la questione con un'interrogazione al Parlamento europeo e nella risposta resa lo scorso 13 marzo la Commissione ha comunicato che è in corso un confronto proprio in tale direzione per ampliare il numero di infrazioni su su cui collaborare in maniera transfrontaliera. A tal proposito, il mio impegno è quello che al prossimo Consiglio europeo dei Ministri dei trasporti previsto a dicembre (la settimana prossima sarò a Budapest per l'interministeriale informale e solleverò il tema sarà portato da me alla luce anche per la recente adozione della direttiva Cross Border Enforcement sull'applicazione transfrontaliera delle infrazioni stradali. Se l'Europa deve dimostrarsi solidale e unita - a proposito di Austria, la chiusura unilaterale del transito al Brennero è un altro tema su cui vogliamo andare fino in fondo *(Applausi)* - questo è uno dei temi su cui lavoreremo.

di un'interrogazione che le avevo indirizzato poco tempo fa, riguardante le società di noleggio che non rispondono più solidalmente con i locatari per le infrazioni stradali e pertanto non forniscono le date. Lei all'epoca mi aveva dato ragione, ma purtroppo, nella sua riforma del codice della strada, non c'è traccia di questo. Si dovrebbe modificare l'articolo 196 e ho predisposto un emendamento,

Signor Presidente, con questa interrogazione ci rivolgiamo al Ministro delle infrastrutture per conoscere le determinazioni riguardo la realizzazione della ciclovia dei due mari, che è un'opera infrastrutturale molto attesa e fondamentale per lo sviluppo del territorio umbro

portando la massa delle persone che si rivolge a questo tipo di turismo lento a occupare veramente tantissimi posti per viaggi e per andare a scoprire angoli del territorio che altrimenti sarebbero rimasti non fruibili.

vorrà tenere presente nella strategicità che ha sottolineato poche ore fa anche l'assessore regionale Enrico Melasecche, che voglio veramente ringraziare per la sua professionalità insieme alla presidente Tesei, che ha fatto di questa grande possibilità di sviluppo del territorio una propria battaglia. L'Umbria è un crocevia degli itinerari ciclabili nazionali. Dall'Umbria passerà la cosiddetta Ciclovia del Sole, un'opera che invece si sviluppa dalla Scandinavia fino alla Sicilia, secondo quello che sarà il progetto poi da realizzare e si interseca con altri tre percorsi, tra cui appunto quello dei due mari, che - guarda caso - attraversano proprio l'Umbria. Quindi vogliamo rivolgerle il quesito per far conoscere la sua risposta agli amministratori umbri che si sono veramente molto distinti rispetto ai predecessori Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Matteo Salvini, risponde all'interrogazione illustrata per tre la realizzazione di una rete nazionale di ciclovie con intermodalità è uno dei primi temi su cui abbiamo lavorato al Ministero. Lo scorso 27 giugno, in sede di Conferenza Stato-Regioni, sul decreto interministeriale che rimodula il programma PNRR ciclovie turistiche in base ai progetti in fase più avanzata abbiamo registrato la richiesta della Regione Umbria e della Provincia autonoma di Bolzano di sviluppare ulteriori piste ciclabili intermodali. intermodali. La Conferenza Stato-Regioni all'unanimità ha dato il proprio assenso al finanziamento di tale opera e il Ministero che sto guidando si è impegnato ad adottare, entro sessanta giorni dalla registrazione del decreto, un provvedimento finalizzato ad assegnare alla Regione Umbria e alla Provincia autonoma di Bolzano le risorse necessarie per la realizzazione di queste ciclovie intermodali. Il decreto interministeriale ciclovie turistiche è ora al vaglio della Corte dei conti; attendiamo la registrazione del provvedimento nelle prossime due settimane. All'esito della pubblicazione del decreto, quindi entro quindici giorni, come Ministero dell'infrastrutture provvederemo a rendere operativi tutti gli investimenti necessari per la realizzazione sia della ciclovia che interessa il territorio della Provincia di Bolzano sia della ciclovia dei due mari, che si vanno ad aggiungere ad altre infrastrutture infrastrutture cicloturistiche in realizzazione in varie Regioni italiane. Con specifico riferimento all'opera richiamata in Umbria, ricordo che la ciclovia collegherà il Mar Tirreno partendo da Grosseto, passando attraverso l'Umbria, fino a raggiungere il Mar Adriatico a Fano, Tale opera si aggiunge alle ulteriori infrastrutture in corso di realizzazione su tutto il territorio umbro: ricordo in particolare i lavori di ampliamento a quattro corsie della statale 318 di Valfabbrica, con l'abbattimento del primo diaframma della galleria Picchiarella, a cui ho partecipato personalmente il mese scorso. Ricordo la realizzazione del nodo di Perugia e le opere ferroviarie che renderanno l'Umbria la cerniera tra Nord e Sud Italia, tra cui la linea Sansepolcro-Perugia-Terni e la Orte-Falconara. L'auspicio è che tali interventi, attesi da tempo, possano consentire un forte aumento di flussi turistici, peraltro già abbondantemente presenti in Umbria, nelle aree interessate dal passaggio della ciclovia turistica. Mi auguro pertanto di poter tornare presto in quest'Aula e sul territorio per informare circa l'avvio dei lavori richiamati dal senatore ripeto, come Ministero e come Governo consideriamo lo sviluppo infrastrutturale del Paese una priorità anche nei territori interni e montani o nelle aree, come quelle dell'Umbria, duramente colpite dai terremoti più recenti. che per troppi anni sono state al margine dei programmi di sviluppo dei Governi nazionali e che oggi, dal mio punto di vista, sono tornate al centro dell'agenda politica per valorizzare un patrimonio storico, artistico, paesaggistico, culturale e sociale di inestimabile valore. Si tratta di finanziamenti concreti e non di meri propositi.

quello strumento che ha un trattamento giuridico deteriore rispetto agli altri veicoli che circolano sulle nostre strade. Devo ricordare - e mi piace elogiarla per questo - le norme che entreranno in vigore in materia di sorpasso di velocipedi e le condizioni per la realizzazione di corsie ciclabili, che finalmente, almeno per quanto riguarda il decreto che il MIT emetterà entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, consentiranno

dimostrato e sta dimostrando di poter portare avanti anche questo importante *asset*, che costituisce un elemento economico fondamentale per i territori.

insieme al mio Capogruppo e a tutti i colleghi di Italia Viva vogliamo anzitutto fare un in bocca al lupo agli studenti che hanno appena iniziato l'anno scolastico e augurare buon lavoro a tutto il personale scolastico. Purtroppo i problemi, Ministro, sono all'ordine del giorno, con un anno che si presenta difficilissimo. Sappiamo che in otto anni - ahimè - è raddoppiato il numero dei precari nella scuola, passando dal 12 per

tutti gli oltre 63.000 posti vacanti disponibili, perché sappiamo che sono previste solo circa 45.124 immissioni di ruolo di insegnanti della scuola d'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, lasciando scoperte quasi 19.000 cattedre. A questi numeri vanno poi aggiunte le decine di migliaia di posti precari, legati soprattutto ai docenti di sostegno. I posti in organico di diritto sono circa 126.000, ma sappiamo che poi in realtà si raddoppiano. Vorremmo sapere dal Ministro quali misure si possano adottare al fine di reclutare un maggior numero di insegnanti e soprattutto stabilizzare un organico di docenti attualmente precari per porre finalmente fine al disastro delle supplenze che ogni anno crea problemi prima di tutto ai nostri studenti, alle famiglie e a tutto il corpo docente. Vorrei inoltre ricordare che proprio oggi l'OCSE che gli insegnanti italiani sono i meno pagati al mondo e che questo Governo destina solo il 4 per cento del PIL all'istruzione. Vorremmo avere in merito delle risposte per il mondo della scuola, ma io dico per tutto il nostro Paese.

mi consente di fare subito chiarezza sul dato OCSE, che si riferisce all'anno scolastico 2021-2022. Quindi, sono dati precedenti al contratto concluso nel 2023 e a quello che si andrà a concludere auspicabilmente nel 2024. Fatta questa premessa, ho già avuto modo di dire che il precariato rappresenta una questione endemica della scuola italiana. Si sono succeduti tanti Governi e nessuno è sinora riuscito a risolvere il problema. Per questo Governo, invece, il tema del precariato è una priorità, come dimostrato dalle azioni di sistema già intraprese che mirano a una progressiva e durevole riduzione del fenomeno. Per comprendere il problema è però prima necessario fare chiarezza su alcuni dati di fatto che sono più forti delle strumentalizzazioni circolate negli ultimi giorni. E mi fa piacere, fra l'altro, che lei non abbia dato credito a dette strumentalizzazioni. Non è vero che attualmente ci sono 250.000 precari nella scuola italiana, come affermato da qualche sindacato e da qualche forza politica. Le supplenze cui dobbiamo ricorrere per coprire l'organico sono infatti pari a 165.000 unità, che si ridurranno a 155.000 entro dicembre grazie alle assunzioni derivanti dai concorsi PNRR che sono in via di chiusura. Quest'anno, dunque, si registrerà già una prima diminuzione del numero dei precari che lo scorso anno e negli anni immediatamente precedenti era pari a 160.000 unità. Quindi a dicembre saranno 155.000 contro 160.000. Va detto anche che la maggior parte dei precari - poco più di 100.000, come d'altro canto riconosciuto anche da alcuni sindacati come CISL e UIL - sono insegnanti di sostegno in massima parte chiamati sui cosiddetti posti in deroga. Per questi posti si rendono disponibili soprattutto docenti privi di specializzazioni; ciò impedisce qualsiasi ipotesi di loro assunzione a tempo indeterminato, proprio perché la legge stabilisce che devono essere assunti in ruolo docenti specializzati sul sostegno. Per questa ragione noi siamo intervenuti alla radice del problema, dal momento che il sistema universitario non si è rivelato adeguato a coprire le esigenze del sistema di istruzione, istituendo di recente nuovi percorsi di specializzazione gestiti da INDIRE, riservati proprio ai docenti precari sul sostegno. Va anche detto che, se quest'anno non abbiamo potuto mettere a disposizione per le assunzioni tutti i 65.000 posti disponibili, ciò discende dal vincolo stabilito dal precedente Governo con la Commissione europea, che ci impone di assumere 70.000 docenti esclusivamente attraverso i nuovi concorsi PNRR. Dunque qualsiasi altra stabilizzazione e qualsiasi altro meccanismo di assunzione non vengano considerati ai fini della *milestone* europea. Fra l'altro, voglio subito aggiungere che questa *milestone*, che dovrà essere realizzata entro il 2026, è collegata alla ultima rata che ammonta a 24 miliardi di euro. Se noi non raggiungiamo questa *milestone*, rischiamo di far perdere al sistema Italia una parte di quei 24 miliardi. anche su tale punto. A fronte di questo obiettivo iniziale oggettivamente irrealistico, siamo riusciti a negoziare una maggiore flessibilità con la Commissione europea, ottenendo una proroga dal 2024 al 2026 del *target* assunzionale. Senza questa flessibilità, non sarebbe stato possibile né bandire il concorso per 46.000 docenti precari appena svolto, né assumere i 6.000 idonei dei precedenti concorsi. A fronte di ciò, però, abbiamo dovuto accantonare circa 19.000 posti per bandire il prossimo concorso PNRR secondo il nuovo *timing* richiestoci dalla Commissione. Insomma, se noi avessimo fatto tutte queste assunzioni, non avremmo potuto non avremmo potuto utilizzare le facoltà assunzionali per arrivare al *target* previsto dalla Commissione. Concludo informando che ho ribadito - anche da ultimo al collega ministro Fitto - la necessità di avere un nuovo confronto con la Commissione europea per ottenere ulteriori margini di flessibilità sulla riforma del reclutamento del PNRR, anche alla luce di una oggettiva analisi della sua prima attuazione, al fine di renderla più aderente alle esigenze concrete del nostro sistema scolastico, favorendo la continuità didattica dei nostri studenti e dando maggiori opportunità ai docenti precari.

questo, Ministro, perché non siamo soddisfatti? Non abbiamo un approccio ideologico - e mi fa piacere che anche lei lo abbia sottolineato - perché questo è il nostro modo di lavorare come Gruppo Italia Viva: essere cioè accanto al Governo quando fa le cose per il Paese ed essere invece all'opposizione in maniera forte e determinata quando si sbaglia. Vorrei aggiungere, Ministro, che, oltre agli insegnanti precari, c'è anche il numero relativo al personale ATA. Parliamo di uno su cinque che è precario e, secondo il dato di analisi relativo al 2023, il 21,64 per cento del personale ha un contratto a tempo determinato. Le ricordo anche in conclusione

dei nostri insegnanti, che fanno un lavoro faticosissimo. Mi avvio a chiudere, Presidente. Più risorse, dobbiamo decidere quali sono le priorità; magari parliamo meno di liceo *made in Italy*, che si è dimostrato un *flop*, oggi fermato anche dal Consiglio di Stato, e parliamo veramente di cose serie.

Pietro Mennea a Città del Messico, nei 200 metri piani, consegnava al nostro Paese un *record* che è rimasto imbattuto per oltre diciassette anni. Era il famoso e mitico 19"72, a dimostrazione di come un ragazzo del Sud, con la sua forza e la sua capacità, in quel

in quest'Aula - è stato anche parlamentare europeo, è giusto ricordarlo. Oggi si fanno tanti eventi durante l'anno, come quest'anno, durante gli europei, è stata coniata la moneta celebrativa. Io mi auguro che, grazie anche alla Fondazione Mennea e alla moglie Manuela Olivieri, si possa avere quanto prima il museo

è importante questo mio intervento, proprio oggi in quest'Aula, per dare voce a quello che sta accadendo sul territorio in quel di Gallarate, in provincia di Varese. Succede che la cittadinanza è in grande fermento, in opposizione alle decisioni del Consiglio comunale guidato dal sindaco Cassani della Lega (se non sbaglio è segretario provinciale della Lega). In pratica stiamo parlando di un progetto di 18 milioni di euro, che va a spostare quattro edifici scolastici ben distribuiti in Gallarate, riunendoli in un nuovo polo scolastico che andrebbe costruito *ex novo* abbattendo un bosco. Allora, considerato che in Gallarate il consumo di suolo arriva al 52 per cento, in netta maggioranza rispetto a quello che accade nei territori limitrofi, l'idea di sacrificare un polmone verde, che tra l'altro fa da cuscinetto con l'autostrada, andandoci a costruire questo mega edificio, è un problema sia dal punto di vista ambientale, sia da quello sociale. Dal punto di vista sociale i cittadini si lamentano, perché i quattro attuali plessi scolastici (stiamo parlando di scuola materna e di scuola elementare) sono ben distribuiti sul territorio, facilmente raggiungibili dalle persone e creano aggregazione. Invece spostare ai limiti della città un unico plesso scolastico crea solo disagi dal punto di vista sociale e dal punto di vista ambientale. Attraverso Legambiente e con il Parco della Valle del Ticino una richiesta al prefetto, che ha svolto un incontro, agli esiti del quale ha chiesto al Comune di valutare la possibilità di ridurre la parte di bosco che viene abbattuta, di evitare gli abbattimenti nel periodo attuale di nidificazione e di monitorare la presenza della fauna selvatica con fototrappole. Tutto ciò è assurdo e paradossale, perché questo viene fatto nell'ottica della transizione ecologica. Dov'è la transizione ecologica nell'abbattimento di un bosco e nel creare una struttura che i cittadini non vogliono? I cittadini peraltro non sono stati interpellati dal sindaco con nessun tipo di partecipazione; il sindaco ha risposto alzando il dito medio. di Pero, che è sempre del ramo di destra, però di altro partito, ha invece deciso di eliminare un progetto similare, sempre di 18 milioni di euro, e di riqualificare l'esistente. C'è da imparare anche tra colleghi di maggioranza.

Grazie